nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e sono stati accantonati gli emendamenti 3.138,

tutti coloro che conoscono il testo degli emendamenti sanno che l'emendamento 3.143 riproduce, in buona parte, nella lettera e totalmente nello spirito, il contenuto di altri emendamenti di cui già abbiamo parlato e tocca il tema fondamentale di cui oggi ci occupiamo, quello della qualificazione giuridica, cioè del nome da dare alla idratazione e all'alimentazione artificiali. Un filosofo del linguaggio francese, Brice Parain, diceva che le parole sono pistole cariche e che se le si maneggia con poca attenzione sparano e possono fare molto male. in questo dibattito e fuori da quest'Aula, le parole hanno sparato parecchio e colpi diretti o di rimbalzo sono andati ad urtare sensibilità e suscettibilità che probabilmente non meritavano. Mi riferisco all'uso di espressioni per sostenere una tesi legittima come «morire di fame e di sete», riferita alla conseguenza dell'interruzione di artificiali procedure per l'idratazione e per l'alimentazione. Mi riferisco all'espressione - non so quanto provocatoria e non so quanto invece nutrita di un'effettiva convinzione - con proprio da lei, Presidente, dagli scranni di senatore, é stato richiesto a chi sosteneva una tesi diversa dalla sua di avere il coraggio di dire che qui si parla di «diritto alla morte». Vede, Presidente, volontariamente - e credo spesso involontariamente - questo tipo di operazioni sulle parole portano a una manipolazione linguistica che produce drammatiche conseguenze sulle coscienze che di questi temi devono occuparsi. La manipolazione delle parole non è mai una buona cosa. Ricordo che - non sono un cattolico praticante, ma trovo che nelle Scritture e, soprattutto, nel Vangelo ci siano grandi insegnamenti per chi è credente, per chi non lo è e per chi ha il suo modo di vedere le cose della fede e della morale - nel Vangelo di Matteo Gesù dice: «Il vostro dire sia sì sì, no no. Il di più viene dal maligno». Qualcuno potrebbe chiedersi cosa c'entra questo con il nostro dibattito; c'entra, perché chiedo: vi sareste e ci saremmo mai posti il problema di dare una così contorta definizione di quelle che pacificamente per tutto il mondo scientifico e legislativo sono pratiche mediche se non avessimo e se non aveste avuto l'esigenza di aggirare una norma costituzionale, anche se la Costituzione non si lascia facilmente aggirare? Questo lo verificheremo, infatti, dopo che questa legge sarà entrata in vigore e dopo che sarà sottoposta a giudizio della Corte, Non vi sareste posti questo problema, così come non vi sareste posti il problema di riflettere - mi sia consentito, senza alcuna intenzione provocatoria - sul concetto di diritto e, in particolare, di disponibilità del diritto in maniera un po' superficiale, quasi che i diritti, ad onta di quello che una riflessione secolare ci ha portato ad apprendere, fossero entità monodimensionali e non, invece, plastiche e complesse entità che acquistano il loro contenuto, il loro significato e la loro forza nel complesso delle relazioni sociali. Un diritto della persona, così come qualsiasi diritto soggettivo, si compone di una serie di sfaccettature, elementi, facoltà, potestà, prerogative di fare, di pretendere e di escludere, signor Presidente. Il diritto all'integrità personale, di cui vi è traccia in tante norme e in particolare in quell'articolo 32 della Costituzione di cui troppo, e forse troppo a sproposito, abbiamo parlato,

voglia penetrare nel suo terreno, che è sua proprietà privata, così il proprietario di un corpo ha il diritto di dire, ora per allora, adesso e in qualsiasi momento, che non vuole che nel suo corpo penetri un oggetto fisico o sostanze

non di un soggetto che ha perso ogni contatto con il mondo esterno. Tale manipolazione linguistica è insopportabile - se mi consentite - perché essa sottende l'attribuzione a chi si attesta su posizioni diverse di un pensiero che non è suo, quasi che da una parte vi sia chi sostiene la vita e dall'altra -

e non ha nulla a che fare con una categoria giuridica del tutto diversa che è la prerogativa di impedire l'invasione di un terreno come del proprio

indefinitamente, in un territorio gelido e desolato che non è vita e non è ancora morte, vogliamo ricordare le ultime parole di un grande Papa, papa Giovanni Paolo II, che disse: «Lasciatemi andare alla casa del Padre».

se ricollegato all'emendamento 3.157, a firma degli stessi proponenti. Esso si colloca nella linea di quegli emendamenti che questa mattina sono stati emendamenti di mediazione o emendamenti ponte. Anche da parte del Gruppo dell'Italia dei Valori vi è il tentativo di rendere questo provvedimento legislativo un provvedimento credibile e, al tempo stesso, sostenibile sul piano della costituzionalità del provvedimento stesso. Questa mattina il senatore Tomassini, con grande onestà intellettuale, ha riferito che la comunità scientifica, con la quale un'Aula parlamentare deve comunque avere un riferimento di dialogo e di interlocuzione, non è unanime nella definizione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiale. Il senatore Astore, con altrettanta competenza, ha riferito che le audizioni, non solo nel

La stessa discussione interessante che vi è stata questa mattina riguardo alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (cioè sul concetto se attenersi o meno all'armonia e non, invece, a quella che sarebbe stata una definizione esatta nell'attuazione della Convenzione) dipende da un aspetto non trascurabile. La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

confronto. La Convenzione, all'articolo 25, richiede agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare ottenendo il consenso libero e informato della persona con disabilità e, quindi, nel rispetto della dignità e dell'autonomia della persona stessa. Questo è quanto dice la Convenzione ONU sui diritti delle persone

di considerarle forme di sostegno vitale qualora, però, finalizzate all'alleviamento della sofferenza umana.

un'alimentazione forzata può acquisire quei caratteri di gravosità, inefficacia ed ostinazione tali

un diverso riconoscimento dei diritti dei cittadini che hanno la capacità di intendere e di volere - quindi la capacità di decidere - rispetto a quelli dei cittadini che questa capacità l'hanno persa, ma che hanno espresso in maniera chiara e

rispetto del diritto di decisione della persona umana è previsto per chi ha capacità di decidere, costituzionalmente non può non essere previsto anche per chi ha perso

lo dico al relatore e ai rappresentanti del Governo - per noi questo è un aspetto di civiltà giuridica, di fondamento giuridico di determinate condizioni della vita.

dice chiaramente che il medico non ha l'obbligo di contrastare e ritardare ad ogni costo l'esito finale della malattia, ma piuttosto, nel rispetto del migliore interesse del paziente, ha il compito di accompagnarlo ed assisterlo verso la sua fine naturale. Questo era quanto dicevano alcuni colleghi del centrodestra sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, sul testamento biologico e dunque sull'oggetto della discussione di oggi.

la PEG o altri non sono più tali, non essendo trattamenti sanitari, quantomeno evitiamo di scrivere che questi trattamenti sanitari non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Nell'ottica della riduzione del danno

segnalo che questo emendamento, come anche quello esaminato nella seduta di ieri, proviene dalla lettera dei filosofi morali di area cattolica che sostengono che, almeno in questi casi, occorre riconoscere la libertà di scelta alla persona. Ne approfitto, inoltre, per replicare su due punti in merito alla costituzionalità. In primo luogo, trovo un po' paradossale l'argomentazione addotta dal collega, senatore Saltamartini, che ha sostenuto che solo una legge rigidamente proibizionista senza se e senza ma sarebbe coerente con la Carta di Nizza. Registro che solo in Italia si sta andando

no. Replico, inoltre, al senatore Nania ed altri, che hanno inventato questa teoria del tutto nuova alla dottrina di distinzione tra diritti inviolabili e diritti fondamentali, che in tutti i manuali si legge che diritti inviolabili e fondamentali sono esattamente la stessa cosa, non c'è distinzione.

Il disegno di legge che stiamo discutendo, lo abbiamo detto tante volte, tocca le coscienze di tutti. L'appello che rivolgo alla maggioranza è di considerare questo emendamento come un testo proposto da esponenti non da esponenti dell'opposizione. Ai colleghi del mio Gruppo chiedo, allo stesso modo, di non guardare a questo emendamento come ad una proposta che viene da esponenti cattolici che hanno come unico desiderio quello di rispondere ad una gerarchia ecclesiastica.

Colleghi, si sta illustrando un emendamento estremamente delicato, al di là della delicatezza dell'intera materia.

Mi rivolgo a tutti voi - almeno ci provo - per permettere all'Aula di svolgere una riflessione profonda, che ci consenta di intervenire con razionalità e umanità su una legge che coinvolge medicina, biologia, vita e morte. La sospensione della nutrizione e dell'idratazione, soprattutto nello stato vegetativo e nei casi in cui un paziente è incapace di intendere e di volere, è inevitabile che generi grandi controversie. Per quanto mi riguarda, non posso non tener conto di alcuni elementi essenziali. Primo: l'individuare la nutrizione e l'idratazione tra gli atti definibili cura o terapia ci permette di richiamare e invocare l'articolo 32 della Costituzione, fondante il principio della libertà di cura. Va detto che i principi costituzionali sono tanti e, gerarchicamente, vanno bilanciati e portati ad un equilibrio giuridico. Pertanto, i principi del diritto alla salute, della solidarietà, della dignità e del rispetto della tutela degli incapaci non possono avere minore avere minore rilevanza rispetto alla libertà di cura. Secondo: deve essere messo in evidenza che la sospensione di idratazione e nutrizione porterà a morte certa ed inevitabile. Appare dunque veramente molto chiara la differenza tra il rifiuto delle cure, a cui si appella l'articolo 32 della Costituzione, e la sospensione della idratazione e della nutrizione. Con il rifiuto della cura il soggetto morirà, probabilmente, a causa della propria patologia, che seguirà il naturale decorso senza l'intervento della medicina. Con la sospensione della idratazione e della nutrizione, invece, il soggetto morirà certamente, non più con la propria patologia, ma per disidratazione e denutrizione. Perché e quando nasce il problema della nutrizione e della idratazione? Nasce nel 1975, quando una giovane di 22 anni, Karen Quinlan, Quinlan, entra in stato vegetativo e i genitori iniziano una battaglia legale per staccare il respiratore che la tiene in vita. Nel momento in cui vincono la battaglia legale e il respiratore viene staccato, l'evento della morte non avviene e quella ragazza continuerà a vivere per altri dieci anni. Altri casi sono quello di Helga Wanglie, nel 1988, o di Baby K, nel 1992. Sono tutti casi in cui viene sospesa una terapia, ma i pazienti continuano a vivere. E allora, colleghi, dico che, mentre questo disattende i principi di inviolabilità della vita, della solidarietà e della intangibile tutela dei soggetti incapaci (princìpi che sono stati fino ad oggi alla base dell'etica medica e della nostra Costituzione, alla quale nessuno di noi vuole rinunciare), va detto altrettanto chiaramente però che la capacità della medicina tecnologica di intervenire nel processo della morte è tale che oggi, in una percentuale elevata di casi, il momento della morte può dipendere soprattutto da una decisione del medico. Quindi, con altrettanta chiarezza e determinazione, va detto che l'idratazione e la nutrizione devono essere sospese nel momento in cui il paziente non è più in grado di assimilare sostanze nutritive ed idratanti perché in questo caso l'idratazione e la nutrizione finirebbero con l'assumere i connotati dell'accanimento terapeutico. Colleghi, il compito del legislatore è quello di definire un limite, di offrire al medico ed al paziente un criterio attraverso il quale poter operare scelte comunque delicate. L'emendamento 3.160 sul quale dobbiamo esprimerci tenta di andare in questa direzione. Per questo chiedo a tutti i colleghi di condividere, con i quattro firmatari, tale emendamento.

grazie. So benissimo che ogni singolo emendamento viene votato in modo autonomo, però chiedo al relatore di valutarli entrambi perché prevedono la stessa identica fattispecie: una unica possibilità di sospensione dell'idratazione e dell'alimentazione qualora si determini un quadro clinico ben preciso e quindi l'accertamento della

- naturalmente, parlo a titolo assolutamente personale - e per associarmi a quanto detto dalle due colleghe che mi hanno preceduto nell'invitare il relatore ed il Governo a considerare a fondo questi due emendamenti che nulla tolgono al significato del comma 6 dell'articolo 3. Sanciscono, infatti,

qualunque terapia può non essere più adatta per il soggetto e può diventare una forma di accanimento terapeutico. Invito pertanto veramente a considerare ciò con grande attenzione perché vi possono essere casi in in cui, non essendoci più assimilazione ed assorbimento, anche l'idratazione e la nutrizione possono diventare accanimento terapeutico.

"La sospensione di idratazione ed alimentazione è possibile solo qualora sia presente evidenza clinica di perdita irreversibile della funzione propria dell'individuo di assorbimento e di metabolismo. La valutazione in merito deve essere formulata dal collegio medico di cui al secondo periodo del comma 7".

il parere del Governo, che è assolutamente conforme a quello testé proposto dal relatore. Siamo, infatti, in presenza di una fattispecie che può riferirsi a quella di un malato terminale la riformulazione del relatore, anche per la collocazione nella quale si verrebbe a trovare all'interno del testo, rappresenta un ovvio, vorrei dire anche opportuno, complemento della definizione principale.

esclude il riferimento, contenuto nell'emendamento Bianchi, comunque al consenso informato ed alla figura del fiduciario. Lei ha cioè

perché delle due l'una: se salta il riferimento al consenso informato si tratta di una direttiva che si dà ai medici, e quindi è una direttiva che solleva dalla responsabilità, si dà una guida, si offre un usbergo ai medici, i quali interrompono l'idratazione e la nutrizione quando l'organismo non sia più in grado di metabolizzarle. Se invece si consente il riferimento al consenso informato, la questione è un'altra: idratazione e nutrizione possono essere oggetto di consenso informato, e quindi di dichiarazione anticipata di trattamento, esclusivamente per quell'ipotesi di fine vita nella quale l'organismo di chi ha dichiarato la propria volontà non sia più in grado di metabolizzare la nutrizione e l'idratazione che gli vengono somministrate. Cambia il senso, questo volevo dire. Cioé, il senso autentico dell'emendamento della senatrice Bianchi viene o non viene tramutato dalla sua riformulazione? noi, signor Presidente. e, in rapporto all'evidenza clinica dei dati che vengono rappresentati in questo emendamento, può fare la scelta della sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione.

l'idratazione e l'alimentazione cessano di essere, "per la contradizion che nol consente", sostegno vitale nei suoi confronti. qualsiasi operatore sanitario che operasse in queste condizioni per idratazione e altro e altro farebbe un'attività inutile che non gli è assolutamente consentita. Ma non gli é consentita non perché è un trattamento sanitario, ma perché non è un sostegno vitale in riferimento al soggetto nei confronti del quale dovrebbe operarsi.

Calabrò - non so se è lui il demonio della frase di San Matteo - che credo non sia possibile introdursi e cercare di dividere gli altri su una questione che noi dobbiamo assolutamente rifiutare. Noi avevamo superato con alcuni emendamenti ponte i termini idratazione e alimentazione, nominalisticamente cioè vi avevamo rinunciato; nostri emendamenti avevano addirittura dichiarato che erano sostegno vitale, ma voi li avete assolutamente rifiutati. Oggi non si può accettare un emendamento

sincero, come lo avevamo impostato nei primi giorni di dibattito in Commissione. Queste furbizie non ci interessano, questi ammiccamenti

*(PD)*. Signor Presidente, annuncio il mio voto decisamente contrario, perché quello che è scritto in questo emendamento significa, con molta chiarezza, lo dice il linguaggio, di assorbire i nutrienti che vengono somministrati. Sarebbe un po' come dire ai medici che dopo diversi tentativi di defibrillare il cuore,

quello che devono fare, lo sanno molto bene e sanno perfettamente che quando il corpo ha cessato le sue funzioni e c'è una situazione di accanimento terapeutico si devono fermare, non dobbiamo dirglielo noi, signor Presidente. Di fronte alla morte non si può che votare contro questo tipo di emendamento.

Quando tutti avranno raggiunto i loro posti e si saranno seduti, la Presidenza valuterà se dare la parola o meno ai colleghi che la stanno votazione. Prima della votazione, avevo pregato il relatore, in un'Aula che potesse ascoltare il senso di quello che si mette in votazione, di ripetere

Presidente, prima di leggere nuovamente la formulazione, il presidente della Commissione intende... PRESIDENTE. No, lei legga per ora la riformulazione. CALABRO', *relatore*. «La sospensione di idratazione ed alimentazione è possibile solo qualora sia presente evidenza clinica di perdita irreversibile della funzione propria dell'individuo di assorbimento e di metabolismo. La valutazione in merito deve essere formulata dal collegio medico di cui al secondo periodo del comma 7".

come questa disposizione sia in qualche modo ultronea, nel senso che si riferisce alla condizione di un malato terminale che rigetta alimentazione e idratazione; potremmo quindi che si produca naturalmente la condizione descritta nel testo, soprattutto nella formulazione del relatore. Il Governo quindi ha condiviso il tentativo di raggiungere un'intesa più ampia, che però sembra non essere possibile; si rimette all'Assemblea per la valutazione che essa riterrà, tanto più che, ripeto, in effetti, questa disposizione probabilmente nulla aggiunge e nulla toglie a ciò che la regolazione complessiva dell'articolo 3 consentirà o meno di fare.

mentre il Governo si sta rimettendo all'Aula, lei, da relatore, ha proposto una riformulazione degli emendamenti 3.160 e 3.161, che costituiscono quindi la sua proposta.

nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico e familiari del paziente o fiduciario. Queste erano le tre condizioni in questo modo, si bilanciava anche quella minima apertura al principio di autodeterminazione, che mi sembrava doveroso vi fosse proprio in quello che era l'articolo più nodale e più delicato di questa legge. Dobbiamo, invece, prendere atto che qualsiasi tentativo serio e vero di dialogo su questo tema non è stato possibile. Devo prendere atto che il dialogo è stato immolato sull'altare della radicalità delle posizioni. Devo prendere atto che non si può andare avanti. Pertanto, l'emendamento 3.162 è ritirato, perché non ha più senso che esista.

Presidente, voglio innanzitutto dire che siamo orgogliosi che, accanto ad una convergenza fondamentale su punti qualificanti di questo disegno di legge

si sia registrata su materie così critiche e complesse l'espressione di un pluralismo effettivo del Gruppo del Partito Democratico. Cari colleghi, penso sia giusto attendersi, all'interno della cornice che si sta formando, che vi siano altre espressioni di libero pluralismo anche nelle file della maggioranza. Sarebbe sufficiente che tutti noi ci ponessimo nell'ottica di leggere questo emendamento come quello il cui contenuto, allo stato - cioè dopo la bocciatura di altri ed il ritiro di qualcun altro possa contribuire per tutti, e non solo per questa o per quella parte politica, ad individuare una sorta di terza via, che non è la negazione delle altre proposte, ma che può essere considerata a cavallo tra una decisione troppo rigida, quale si sta venendo venendo a conformare e quale sarebbe quella prescritta da questo disegno di legge, se venisse così approvato, e una che avrebbe voluto imporre comunque di rispettare la volontà dettata dal soggetto. Con l'emendamento 3.163 si prevede che, nel dialogo forte con familiari e fiduciario, è al medico - tenuto conto di tutto ciò che ci siamo detti - che deve spettare l'ultima parola. sulle fasi terminali della vita e non solo sugli stati vegetativi: in questo modo si approfondisce e si valorizza il dialogo virtuoso tra la volontà del soggetto, l'eventuale fiduciario, i familiari e il medico curante.

che, a nostro avviso, può soltanto nuocere gravemente all'efficacia di questa legge. È una legge che attualmente, da come si va componendo alla luce dell'approvazione di alcuni precisi emendamenti voluti dalla maggioranza,

oltretutto affatto rassicuranti per la tenuta della normativa che stiamo per licenziare. Durante i lavori di questa mattina, il senatore Gasparri ha citato, come presidio della posizione del suo Gruppo, tre passaggi della legge che tutelano i cittadini rispetto all'accanimento terapeutico. Vede, presidente Gasparri, tutti i tre punti da lei citati sono stati rimossi con emendamenti proprio nella mattinata di oggi:

le chiediamo dunque quale preoccupazione ulteriore residui, da una parte e dell'altra di questo Senato, nell'accogliere, dopo che sono state bocciate tutte le altre proposte di modifica, quest'ultima soluzione ponte.

di non cristallizzare le contrapposizioni, dando al Paese la sostanza di una classe politica che su queste materie non ragiona con spirito di parte, ma nell'interesse dei cittadini, la cui vita quotidiana

quest'ultima possibilità, con lo spirito di chi vuole concorrere a realizzare la migliore legge possibile nelle condizioni date

il medico curante decide commisurando la loro modulazione e la via di somministrazione alle condizioni del paziente, non dando corso ad accanimento terapeutico e avendo cura di dialogare con l'eventuale fiduciario e i familiari». Ma anche se il paziente è cosciente? Cioè, ma il medico decide da solo o con un familiare. E il paziente? Il paziente non c'è più.

Forse va riformulato, forse non volevate dire questo, ma vi prego fate attenzione. Presidente Bonino, ho già detto, alla fine del mio intervento, che stiamo cercando delle soluzioni e, siccome quest'Aula ha bocciato tutte le altre soluzioni, dopo questa soluzione c'è solo quella soluzione. Va bene

per cui mi sembra assolutamente scontato che sia assente il paziente ma sia richiamata la presenza del fiduciario.

Questa è l'attività quotidiana dei medici. Se non lo ribadiamo, siccome non è contenuto nel principio di accanimento terapeutico perché è stato cancellato nella legge ogni riferimento all'obiettivo di cura e di sostegno, si apre, secondo me, un equivoco grave per cui si intende che l'interruzione non è mai possibile. E invece sappiamo che non è vero perché nella pratica clinica questo non è.

Prima di proseguire, informo l'Aula che, per consentire ai Capigruppo di partecipare alla Conferenza dei Capigruppo convocata per le ore 20, i lavori d'Aula di questa sera si concluderanno per quell'orario.

testo. Il modo con cui io intenderei riformularlo lo rende lievemente più semplice: esso sarà composto soltanto da un neurologo, da uno psichiatra e da un medico specializzato nella patologia di quella persona. immaginiamo che per applicare una legge dobbiamo chiamare un consesso di cinque superspecialisti, tra cui un neuroradiologo con competenza certificata nella lettura di immagini di neuroradiologia,

con un'organizzazione speciale sul territorio, affinché vengano nel momento in cui si deve prendere la decisione. Io credo che già avere tre specialisti (un neurologo, uno psichiatra e un medico specialista nella patologia in oggetto) possa essere più che sufficiente; questa è la ragione per cui chiedo la votazione di questo emendamento.

Presidente, non vorrei essere pedante, ma c'è un collega che non è presente in Aula e che ha lasciato un fermo

e si diceva tra l'altro che non sono più in grado di intendere e di volere, quando appare tautologico che nello stato vegetativo non si è in grado di intendere e di volere. Con questa riformulazione ampliamo leggermente l'applicazione ai pazienti in coma, che sono in assenza di coscienza e delle funzioni somatiche (peraltro una dizione neurologica un po' desueta, tratta da qualche manuale)

delle aule di tribunale, voglio chiedere se in questa dizione per esempio sono compresi i pazienti con malattia di Alzheimer o pazienti che non sono più capaci di intendere e di volere per grave patologia psichiatrica. Vorrei un chiarimento

appare sempre più chiaro che questa legge ha un contenuto astratto e filosofico, ma che non avrà nessuna implicazione nella vita reale, anzi complicherà molto la vita nelle nostre corsie, nei nostri ospedali e per i nostri cittadini.

in quanto estende l'opportunità di utilizzare la DAT non solo ai pazienti in stato vegetativo ma anche ai pazienti in stato di assenza di coscienza. Voglio sottolineare

Signor Presidente,

alla vita. La formulazione che il relatore e il proponente Malan ci formalizzano aprirebbe allora ad una casistica di persone che invece vanno assolutamente protette e curate (anche pesantemente, vorrei quasi dire), perché c'è ancora la possibilità di tornare indietro, di tornare alla vita. Tra l'altro, Presidente, ripeto ancora una volta: questa norma non la interpretiamo noi e non la interpretano i medici, ma la potrebbero interpretare

e lo stesso relatore con il suo testo base, aveva chiesto di blindare.

Come vedete, ragazzi, il Senato lavora a pieno ritmo.

Non chiarisce però le perplessità che avevo sollevato io. Cosa c'entra la Convenzione dei disabili con i soggetti incapaci? Qui stiamo sovrapponendo due concetti in maniera pericolosissima: si

era soppressivo, senatore Lusi.

la cancellazione, dunque viene precluso.

parteggiando apertamente addirittura per alcune parti della stessa maggioranza. dalla senatrice Bianchi, non era per mettere insieme l'Assemblea, per discutere tutti insieme, ma per mettere insieme una parte di quest'Assemblea. non è così. Le posso assicurare che la Presidenza aveva interrotto i lavori d'Aula anche durante la mattinata perché non vi erano i presupposti per poter discutere. Avevo chiesto al relatore di leggere all'Aula quello che si stava votando, ma non vi erano le condizioni di uditorio tale da far comprendere ai senatori cosa si stava votando e ho sospeso la seduta. Lungi da me l'idea di consentire a qualcuno

quando le interruzioni servono a determinate cose. Comunque, avremmo preferito che lei ne facesse cento di sospensioni, pur di andare ad una buona sintesi su questa legge. L'articolo 3, che è centrale e di cui abbiamo tanto parlato, si pone nel solco di un peggioramento continuo di questa legge. Gli stessi emendamenti approvati, le stesse modifiche fatte non sono altro che peggiorative, signor relatore. Per esempio, cancellare

Esprime una volontà, credo; non può dare un orientamento, altrimenti decide qualche altra persona. Questa legge è così, deciderà qualche altra persona. Avete cancellato il comma 3,

studiate a tavolino da qualcuno per poter peggiorare una legge che era già pessima all'inizio.

al comma 6 e cosa succede? L'Aula lo cancella. Questo mi pare che sia il massimo di chi vuole assolutamente andare verso il peggioramento di questa legge. Parlo dell'emendamento presentato

da chi parlava di libertà personale? Ma è possibile che una legge dia a chi è in vita la possibilità di rifiutare tutto a chi invece è nelle condizioni di stato vegetativo di non rifiutare niente? Mi sembra veramente una sproporzione, una contraddizione nei termini. È questo che volevamo con la legge? Sono in vita, vado in ospedale,

Invece, la mediazione poteva essere veramente ottenuta su questo aspetto, perché quell'alleanza terapeutica di cui vi abbiamo tante volte parlato serve anche a certe convinzioni e a modificare determinate cose. Vi erano anche emendamenti

titolo personale. Il mio dissenso è molto limitato, perché chiedo di non partecipare al voto in quanto la mia contrarietà alle DAT è assolutamente risaputa,

Presidente, ieri abbiamo già compiuto dei passi importanti e mi preoccupa il fatto che nell'agitazione di un dibattito vissuto con passione possano sfuggirci i passi rilevanti che a mio avviso

abbiamo creato le premesse e il fondamento di una legge che fosse rispettosa della Costituzione e laica. Il senatore Maritati ha ripetuto quest'oggi, a proposito dell'articolo 3, l'intervento da lui compiuto già oggi in Commissione Sanità:

Questa è una legge laica, libera, che nel Parlamento trova la sua sublimazione nel rispetto delle norme fondanti. Non abbiamo seguito i *diktat* di nessuno, abbiamo lavorato insieme e - ripeto

non con compromessi, ma con le giuste mediazioni che potessero al meglio interpretare il rapporto tra la norma costituzionale, e l'intendimento, il proposito con cui giungevamo a questa legge. Questo è uno degli elementi più importanti da tenere presente. altro dato di rilievo è che ieri sera noi abbiamo concluso l'approvazione del consenso informato: una novità assoluta nella nostra legislazione, un momento di chiarezza e di tutela del paziente, un momento che dà la libertà al paziente di potersi interfacciare con il medico e con il rapporto dello Stato nella prestazione delle cure e delle attenzioni e, certamente, un momento di grande rilievo. Oggi abbiamo affrontato un altro dei quattro capisaldi di questa legislazione che è, esattamente, quello del contenuto e dei limiti della DAT e soprattutto, nello specifico, ciò che riguarda l'idratazione e l'alimentazione.

quest'Aula, con voto più ampio della maggioranza politica, ha convenuto che l'idratazione e l'alimentazione sono un sostegno vitale da tenere fino alla fine della vita. Questo è il risultato maggiore di questo articolo ed è un risultato condiviso, presidente Finocchiaro. L'emendamento della presidente Finocchiaro, infatti, riconosceva questo fatto. L'emendamento che rappresentava in modo maggiore il Gruppo dell'opposizione, nella sua prima parte, senatore Zanda, è assolutamente identico all'espressione che io sto usando: è sostegno vitale fino alla fine della vita

la conquista importante di questo momento di legislazione. Il relatore ha avuto la capacità, la pazienza, la forza di ricercare soluzioni in qualche modo condivise. Non avevamo forse anche in Commissione, senatore Bosone, senatore Marino, cercato tutti il limite,

avevamo tutti scelto la strada di cercare, in un confronto di scienza e di coscienza, la possibilità incognita che questo *quid* potesse esservi. Questo è stato il tentativo compiuto, anche quest'oggi in quest'Aula, da parte del senatore Calabrò e del Governo ad opera del ministro Sacconi.

L'Aula non può trovare, attraverso le coordinate scientifiche, la forza di promuovere una scelta di tipo politico-istituzionale. La scienza deve fare il suo lavoro e noi dobbiamo dare gli indirizzi con quella serenità con cui un'Aula legislativa attenta è in grado di operare. Io vorrei che qualcuno confrontasse il primo testo inviato in Commissione da parte del senatore Calabrò con ciò che ne è uscito oggi. Quanti passi, senatore Astore, sono stati compiuti insieme. Quanto diverso è il ruolo, più pregnante e presente del fiduciario. quanta chiarezza si è cercato d'intervenire, sia pure su scelte non condivise e che però diventano chiare, su ciò che una parte ha proposto e una parte ha deciso di rigettare. Molto più chiaro, però, in questa definizione è il testo, signor Presidente, che in questo giorno l'Aula ha affrontato. Lo dico per la serenità di tutti e per l'affermazione di un ruolo alto

fatto naturalmente per difendere un interesse di casta, mentre chi avesse votato a favore, sarebbe stato per la vita e per l'ascolto dei cittadini che sono al di fuori di quest'Aula. Su tratta di un'affermazione grave, che non può certamente rappresentare lo spirito di nessun senatore seduto in quest'Aula, né da un parte,

che abbiamo voluto realizzare e di un impegno che abbiamo voluto rispettare.

ad un punto cruciale di questa legge. Devo dire, con grande rammarico, che si era partiti con una certa volontà nella passata legislatura,

da quello che in questo momento stiamo portando al voto articolo per articolo. Avevamo un compito che secondo me - non voglio minimizzarlo - era relativamente semplice: quello di rendere attuale un principio già molto ben scritto nell'articolo 32 della Costituzione. Erano cambiati i tempi: la Costituzione è stata scritta nel 1947, prima che esistesse molta della tecnologia disponibile. Come ho detto tante volte (ma lo voglio ricordare ancora), il primo respiratore automatico è stato inventato nel 1952, la nutrizione artificiale alla fine degli anni Sessanta. Insomma,

del quale mi rammarico molto, perché non credo che alla perdita della coscienza debba corrispondere la perdita dei diritti.

«Valutando che il diritto di autodeterminazione non dovrebbe perdersi semplicemente perché un individuo è incapace di percepire una violazione di esso, questa Corte ritiene che individui incoscienti conservino il diritto di rifiutare un trattamento. Noi riteniamo altresì che tale diritto possa essere esercitato da un decisore sostituivo, quando vi è prova chiara che la persona incosciente lo avrebbe esercitato. In nessun caso può essere costituzionalmente accettabile»

I componenti di una famiglia sono meglio qualificati a dare giudizi sostitutivi per pazienti incoscienti, non solo in ragione della loro particolare capacità di comprendere l'approccio del paziente alla vita, ma anche in ragione del loro speciale legame con lui o con lei. Lo Stato, al contrario, è uno straniero per il paziente. Nessuna distinzione materiale» - e qui vado al punto relativo alla nutrizione all'idratazione e qualsiasi altro trattamento medico. La somministrazione artificiale di cibo e acqua è considerata trattamento medico dalla professione medica e dalle società scientifiche». Questo punto è stato sottolineato con molta chiarezza in quest'Aula, in questi giorni, dal professor Veronesi ed è stato sottolineato da tanti appartenenti alla classe medica.

fare un'incisione nell' addome di una persona, introdurre una cannula, mettere dei punti chirurgici richiede la partecipazione di un anestesista, di un chirurgo, di un gastroenterologo, di un nutrizionista. Ma vogliamo davvero prenderci in giro e dire che questi non sono trattamenti sanitari?

che se occorre un intervento chirurgico quello deve essere definito trattamento sanitario e neanche su quel punto siamo stati capaci di trovare un accordo.

alle persone più care che, se si trovasse in quelle condizioni, non vorrebbe essere portato in una sala operatoria e sottoposto alla introduzione chirurgica di una cannula per la nutrizione artificiale, mentre i medici, dopo avergli detto «questa è la legge dello Stato, lo devo fare», lo porteranno contro la volontà espressa in precedenza e contro la volontà espressa dai familiari in una sala operatoria. Cosa farebbero le persone in quest'Aula se si trovassero in quella condizione? Lo sappiamo tutti cosa farebbero: si rivolgerebbero al magistrato, ed è questo ciò che accadrà! Stiamo scrivendo una legge confusa, una legge che non aiuterà i nostri cittadini,

Concludo annunciando che il Partito Democratico voterà decisamente contro. Il Partito Democratico si pone dei dubbi, lo abbiamo visto, e questi dubbi costituiscono una ricchezza per il nostro Partito, almeno noi la consideriamo tale. Consideriamo il fatto

Aggiungo che la vera differenza tra noi e questa destra è che noi di fronte alla sofferenza riflettiamo, pensiamo e invece questa destra sembra conosca sempre le risposte giuste ad ogni domanda.

il Senato approva

Colleghi, c'è un problema di serietà. Lasciate stare il relatore, che deve ascoltare l'illustrazione degli emendamenti, almeno come atto di cortesia istituzionale.

a prendere atto che dei trattamenti medici, dei trattamenti sanitari, dei veri e propri interventi chirurgici... Ebbene, un'intera giornata non è bastata a sollevare l'attenzione del relatore e della maggioranza su quella che è la realtà fuori da quest'Aula. Quindi potremmo stata spesa inutilmente, nel certificare ciò che qui dentro abbiamo deciso di chiamare con un nome, sostegno vitale,

L'articolo 4 tratta della forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento.

accettati gli emendamenti in cui, invece che il medico di medicina generale, si propone il medico di fiducia. Temo altresì che non saranno migliorate nella loro durata, perché comunque sarà l'unico testamento che avrà un termine, a differenza degli altri testamenti che ciascuno può liberamente redigere e che non hanno scadenza; invece, le dichiarazioni anticipate di trattamento potranno essere valide soltanto per cinque anni e poi bisognerà sottoporre nuovamente il tutto ad un medico che le deve perfino sottoscrivere. Il mio timore è che di queste dichiarazioni anticipate di trattamento che, come abbiamo scritto in Commissione, sono vincolanti,

dannosa, per certi versi, e inutile, per altri. L'esserci sottoposti a queste giornate intere passate in

che parte da una scelta per quanto riguarda le dichiarazioni anticipate di trattamento, le DAT. Esso muove da una considerazione che si fonda sulla eccezionalità, sulla straordinarietà e peculiarità di queste dichiarazioni, sul loro ruolo assolutamente singolare e quindi sulla necessità che la dichiarazione anticipata di trattamento sia rivestita di una forma rigorosa.

di abitudine, debbano essere solenni: e la solennità è data da un certo tipo di forma. Lo stesso però, Presidente e colleghi, non si può dire per la revoca, perché essa può essere manifestata anche in forma libera, verbale, senza l'assistenza del medico, senza cioè quel ritualismo che in queste dichiarazioni

della dichiarazione dai vincoli formali. Dev'essere una revoca espressa, chiara, netta, non contestabile, ma può essere anche formulata in maniera non formalistica come, invece, avviene per la dichiarazione anticipata di trattamento. Quindi, questo emendamento ha tale finalità e mi sembra rientri pienamente nella logica del sistema, laddove si faccia quella scelta

esercitare la propria libertà; non sono neanche vincolanti, perché il medico potrà tenerne conto e potrà seguire alcune indicazioni, ma esse dovranno sempre essere rivolte al benessere ed al meglio per il paziente, seguendo la deontologia.

Proprio perché la parola "vincolanti" introduce un dibattito non sempre chiaro e proprio perché riteniamo di rispettare la libertà e la volontà

Signor Presidente, affronterò soltanto due questioni relative a due emendamenti. La prima fa riferimento all'emendamento 4.23 e riguarda uno dei punti fondamentali di questo disegno di legge: la vincolatività.

rilevo che con tale emendamento andiamo in un senso esattamente contrario rispetto a quanto indicato dalla senatrice Bianconi.

Ricordo che all'interno della Commissione giustizia, come Partito Democratico, avevamo proposto di inserire nel parere di merito, come vincolo per la Commissione sanità, la natura vincolante di tali dichiarazioni anticipate.

«sono vincolanti», si fa subito riferimento all'articolo 7, che parla invece di possibilità per il medico di disattendere le dichiarazioni anticipate del paziente. Quindi, è una contraddizione in termini, che non è assolutamente accettabile.

comma esclude l'utilizzo della dichiarazione anticipata di trattamento quando si versi in condizioni di urgenza. È un'indicazione generale che, a mio parere, non ha alcun senso perché la situazione d'urgenza può benissimo essere indicata

Per questi semplici e banali motivi le chiedo la cortesia di voler sollecitare il Ministro competente a rispondere entro le prossime ore in Aula a quest'importante interrogazione.

fa in relazione ai risparmiatori che hanno avuto la sfortunata ventura di avere nel loro pacchetto obbligazionario

Conseguentemente chiedono - e credo che in questo siano corretti nel farlo - che il loro investimento venga equiparato al normale risparmio che si fa e che abbiano le tutele che il risparmio ha anche costituzionalmente. Le proposte che avanzano sono state da me sottoposte al Ministro. Credo Credo che sia corretto in questa situazione quantomeno fornire una risposta, che certo mi auspico positiva.

nuova finestra") che ho presentato, per la verità, non molto tempo fa, ma che purtroppo assurge a motivo di urgenza per una casualità che non dipende dall'Aula.

Da nove anni si dichiara innocente e in questi giorni sta portando avanti, assieme ai suoi avvocati, quella che forse potrebbe essere la sua ultima possibile istanza, vale a dire un ricorso alla Corte federale.

hanno già sottoscritto questa interrogazione per darvi maggior forza. Il termine l'ho dovuto chiudere per presentarla con urgenza, ma se qualcuno volesse ancora dare come segno di solidarietà

Presidente, intervengono relativamente ad alcune proposte di legge che sono state depositate in 6a Commissione. Il Senato è stata distratto dai lavori non proficui sul testamento biologico. relativi alla garanzia sovrana che l'Italia si dovrebbe assumere nei confronti degli italiani espulsi dalla Libia vent'anni or sono e che vantano dei crediti nei confronti del Governo libico anche a seguito delle espropriazioni. Oggi, il presidente della Camera Fini ha detto che era doveroso, per quanto riguardava l'Italia, chiudere con il proprio passato coloniale. All'interno di questo passato coloniale, oltre alle violazioni dei diritti umani subite dai libici per opera di due regimi con i quali non abbiamo molto a che fare (il fascismo e il Regno d'Italia), molto probabilmente bisogna prendere in considerazione le legittime e altrettanto documentate, checché se ne dica, richieste di alcune migliaia di imprese italiane. Sono delle cifre che in parte già il ministro Frattini diede per coperte quando se ne discusse nel mese di ottobre proprio in Commissione finanze.

molto probabilmente si riuscirà, anche tramite audizioni o iniziative straordinarie, a far emergere la documentazione che ancora oggi non è stata prodotta o a trovare una soluzione che, comunque,

dopodiché, come lei sa, i lavori della Commissione e le priorità con cui affronterà i vari argomenti sono frutto delle decisioni autonome che la Commissione stessa prende come Presidenza e come rappresentanti dei vari Gruppi. Comunque, la sua sollecitazione in Aula è stata registrata. Senatore Di Giovan Paolo,